L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

non possiamo non ricordare come ad esso corrispondano quasi sessantaquattro anni di ininterrotta appartenenza alle Assemblee parlamentari, dalla Consulta Nazionale all'attuale XVI legislatura repubblicana. Buona parte di questi anni sono stati vissuti ricoprendo rilevanti incarichi di Governo: salvo alcune eccezioni, infatti, tutti i Governi della Repubblica, fino al 1992, hanno visto il presidente Andreotti fra i loro membri, per ben sette volte con il ruolo di Presidente del Consiglio. Meno noti, ma altrettanto importanti, gli incarichi di responsabilità ricoperti dal nostro collega all'interno del Parlamento. Nel corso della V legislatura, venne eletto Presidente del Gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana alla Camera dei deputati, nel momento in cui i nuovi Regolamenti parlamentari, approvati nel 1971, cominciavano ad attribuire ai Gruppi, ed in particolare ai loro Presidenti, un ruolo fondamentale nella vita delle Assemblee. Per l'intera durata dell'VIII legislatura, è stato poi Presidente della Commissione affari esteri, sempre presso la Camera dei deputati, in un periodo assai delicato sul piano delle relazioni europee e mediterranee, nel quale iniziava a muovere i primi passi lo strumento della cosiddetta diplomazia parlamentare, al cui sviluppo ha certamente contribuito poi nel ruolo di Presidente della Commissione affari politici e disarmo dell'Unione interparlamentare. A tal punto egli è stato un protagonista della vita pubblica del nostro Paese, che numerosi tratti della sua lunga ed intensa biografia si sovrappongono, quasi confondendosi, ad altrettanti fondamentali momenti e periodi della nostra storia nazionale. La passione politica non esaurisce affatto, però, la complessità e la ricchezza della sua personalità. A questa si affianca, ad esempio, una tenace passione per la scrittura. Avviatosi giovanissimo all'attività giornalistica, ha diretto il periodico della Federazione degli universitari cattolici italiani «Azione Fucina» e successivamente ha continuato ad alternare ai suoi incarichi pubblici una intensa e curatissima attività editoriale. Hanno visto così la luce veri e propri gioielli di analisi storica, trattati con stile lucido e serrato ma sempre aperto alla comprensione dei non professionisti, insieme ad una ineguagliata produzione di memorie e commenti, che ci offrono la preziosa testimonianza di un protagonista dei principali avvenimenti della vita del nostro Paese. Questa sua duplice natura, di uomo politico e di uomo di lettere, ha ricevuto la sua più importante sanzione nel 1991, quando il presidente della Repubblica Cossiga lo ha nominato senatore a vita per altissimi meriti in campo sociale e letterario: lasciò quindi l'Aula di Montecitorio, dove sedeva sin dai tempi della Consulta Nazionale, per entrare a far parte della nostra Assemblea. La sua azione, nei diversi ruoli ricoperti fino ad oggi, è sempre stata animata da una ferma convinzione della centralità dell'Istituzione parlamentare nella vita pubblica. Questa impronta si è sempre manifestata in tutti i suoi atti, sia come parlamentare che come uomo di Governo. II suo profondo rispetto nei confronti del Parlamento si manifesta, inoltre, con l'assidua presenza ed attenzione con la quale egli partecipa, ancora oggi, ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti. I suoi interventi, sempre sagaci nello spirito quanto misurati nei toni e ricchi di saggezza ed esperienza, costituiscono di frequente una pausa di approfondimento e riflessione che cattura l'attenzione dell'intera Assemblea. La matrice profondamente cristiana della sua coscienza di uomo e di cittadino, sempre apertamente rivendicata come tratto essenziale della sua identità politica, traspare anche nella grande sensibilità ed attenzione manifestate nei confronti degli strumenti pubblici di attenuazione delle disuguaglianze sociali nonché nell'intensa ed efficace attività svolta negli anni dalle diverse istituzioni private da lui dirette od animate. È il caso, ad esempio, delle associazioni rivolte a sostenere, mediante sovvenzioni di varia natura, il progresso negli studi di ragazzi "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" (secondo la formula della nostra Costituzione),

un insegnamento prezioso: la sua continua ricerca di un rapporto con i cittadini, anche al di là di quello che è comprensibile e naturale per qualsiasi uomo politico. Una relazione assidua, in grado di esprimere interesse ed attenzione nei confronti della vita, dei bisogni, delle aspirazioni delle persone, e di farsi strumento di una convinta, costante ricerca di autenticità nell'esercizio della rappresentanza politica

oggi compie novant'anni un grande protagonista della politica e della vita democratica del nostro Paese. I senatori dell'UDC, SVP e Autonomie, Gruppo parlamentare che si onora di averlo come collega, formulano i più affettuosi auguri di compleanno al senatore a vita Giulio Andreotti. Andreotti. Con così poco tempo a disposizione, come si può ripercorrere, senza incappare in qualche vistosa dimenticanza, le tappe che hanno reso Giulio Andreotti il grande campione della politica italiana?

Dal 1948, cioè da quando l'Italia è diventata una Repubblica, Giulio Andreotti è stato sempre presente nella vita istituzionale del Paese. Le sue qualità politiche sono note a tutti: pragmatismo, intuito, forza delle idee, lucidità e semplicità, capacità messo a servizio dei cittadini. Il tutto condito da una punta di ironia, la stessa con cui si è sempre divertito a stuzzicare la stampa e l'opinione pubblica, che gli ha affibbiato i più disparati soprannomi e nomignoli, spesso ingenerosi. Giulio Andreotti è l'uomo politico che ha contribuito in maniera determinante alla costruzione del più importante partito del dopoguerra, la Democrazia Cristiana. La sua preziosa militanza nella DC, della quale non assunse mai la carica di segretario, è stata quella del politico puro, rigorosamente e orgogliosamente di professione, che ha sempre inteso la politica come un'arte nobile, come una cosa seria che non si può in alcun modo improvvisare, e che ha sempre diffidato della categoria dei cosiddetti prestati alla politica. La politica italiana e internazionale l'ha sempre visto protagonista; dal periodo della ricostruzione degasperiana alla nascita del Governo di solidarietà nazionale, che nel 1978 aiutò l'Italia ad uscire dal periodo più buio della sua storia democratica. sua capacità e la sua esperienza nel gestire i grandi eventi di politica internazionale, anche i più drammatici, che hanno contraddistinto il dopoguerra? Specie per noi, parlamentari dell'UDC, poi, Giulio Andreotti rappresenta un modello, in particolare, per com'è riuscito in tanti anni a coordinare le sue cariche con il rispetto dei valori cristiani e della funzione della Chiesa cattolica. Un punto di riferimento irrinunciabile, insomma, per l'azione politica nostra, ma anche di molti rappresentanti di partiti di maggioranza e di opposizione che siedono in quest'Aula. Nel corso degli innumerevoli incarichi ricoperti ha sempre mantenuto altissimo il suo senso dello Stato: non ha mai dato peso, forte della verità, alle critiche ed alle accuse che gli sono piovute addosso in tanti anni di Governo. È un uomo dello Stato e, come tale, si è sempre comportato, dimostrando fiducia nelle istituzioni, anche quando le stesse sono apparse ingiuste e ingenerose nei suoi confronti. Mai Andreotti - è bene ricordarlo - ha cercato scappatoie e sotterfugi per evitare il giudizio della magistratura, quale ha sempre dimostrato rispetto e fiducia, anche quando sembrava non meritarlo, ed è stato ricambiato - seppur dopo molto, troppo tempo - con il riconoscimento della verità dei fatti. A partire da questa legislatura - lo ricordo - è componente, da senatore a vita, del Gruppo che ho l'onore di presiedere: da parte nostra, quindi, assieme agli auguri, si rinnova il sentito ringraziamento per l'attenzione che ci riserva e, in modo particolare, gli giunge un ringraziamento da parte degli amici altoatesini, che vogliono riconoscere e ricordare il suo impegno per i problemi del Sud Tirolo e delle sue prerogative speciali. Ancora oggi, si guarda giustamente, con profonda ammirazione e rinnovata curiosità, alla figura di Andreotti. L'Italia, nel celebrare i suoi 90 anni, prova ancora a carpirne i segreti di una vita, spulciando i suoi archivi, cercando interpretazioni sempre nuove alle sue parole e alle sue attività, a ciò che ha contribuito a renderlo unico. Fiumi di inchiostro sono stati spesi per delineare il suo profilo: è stato imitato, oggetto di film, libri, canzoni. È stato, in sostanza, capace di far discutere e appassionare intere generazioni alla politica, ma per tutti noi Giulio Andreotti è soprattutto un padre della democrazia, un patrimonio che il resto del mondo ci invidia, uno scrigno che racchiude, con ordine e cura, un tesoro inestimabile, rappresentato da 60 anni di storia italiana. Signor Presidente, mi consentirà una battuta di spirito affettuosa nei confronti del Presidente del Consiglio, sappiamo - da tempo è alla ricerca del segreto della longevità politica: penso che un paio di consulti con il nostro presidente Andreotti potrebbero essergli molto utili. Al senatore Giulio Andreotti rivolgiamo, con affetto, tantissimi auguri di cuore.

Signor Presidente, l'augurio al senatore Giulio Andreotti è il riconoscimento ad una vita spesa per la famiglia e la politica di questo Paese. Un'esperienza, la sua, cominciata da giovanissimo, accanto ad Alcide De Gasperi, e che ha attraversato tutte le vicende del dopoguerra. Uomo di Governo come nessun altro, ha avuto luci ed ombre, specie nell'ultima parte della sua vita politica, nella quale ha dovuto subire un processo con accuse pesanti, da cui è uscito e di cui ci restano il coraggio e la dignità con le quali ha affrontato il tutto. Si possono non condividere molte delle sue scelte, come ad esempio la sua visione centralista dello Stato l'essere stato protagonista attivo della politica della prima Repubblica, e credo, per quanto ci riguarda, che ben pochi siano stati i punti di incontro tra lui e il movimento della Lega Nord. occorre altresì riconoscere la sua capacità di guidare il Paese con fermezza in alcuni suoi passaggi drammatici, come quelli succeduti al rapimento dell'onorevole Aldo Moro, così come va riconosciuto il suo prestigio internazionale. Come ha recentemente ricordato il senatore Francesco Cossiga, egli è stato una sorta di Segretario di Stato della Chiesa, poiché è sempre stato il ponte politico oltre il Tevere, l'interprete più autorevole degli indirizzi del Vaticano. Anche a noi della Lega Nord farebbe piacere - come le è già stato augurato dalla nostra vice presidente del Senato Rosi Mauro - che potesse dedicare ancora parte del suo tempo allo studio della marineria padana veneziana, che è stata baluardo contro l'invasione dell'Islam verso l'Europa cristiana, così come ha ben fatto con lo studio sulla marineria pontificia. Andreotti occorre sottolineare anche il rigore personale e l'intelligenza politica, non disgiunta da una capacità infaticabile di seguire la vita parlamentare in una carriera che lo ha visto ricoprire tutte le più alte cariche dello Stato ad eccezione del Quirinale. Oggi è ancora una vivace e acuta presenza nel Parlamento e nel Paese e, soprattutto, la formidabile memoria storica della nostra Repubblica uscita dalla lotta di Liberazione. Lunga vita al senatore Andreotti e l'augurio che possa continuare nell'esercizio di quella disciplina politica che è stata la passione e la ragione della sua vita.

Signor Presidente, auguri al presidente Andreotti. Molte parole sono state dette e scritte su Giulio Andreotti nel tempo e, soprattutto, in questi giorni che accompagnano il suo novantesimo compleanno: storici, scrittori, giornalisti, storici, uomini di cultura, di Chiesa e delle istituzioni hanno ricordato e narrato - a volte in termini generosi a volte no - alcuni aspetti della sua storia personale e politica che hanno segnato un'epoca. Mi sarebbe piaciuto anche narrarvi alcuni aneddoti personali, perché Andreotti è stato il mio Presidente del Consiglio quando ero Sottosegretario, il mio Presidente all'Unione interparlamentare e abbiamo anche pregato insieme, ma il luogo e la circostanza esigono una formale e meritata modalità di intervento. Perciò, anche andando un po' fuori dagli schemi di circostanza, desidero accompagnare l'augurio di tutto il Gruppo del Partito Democratico del Senato - ma credo di poter dire di tutti i senatori, come ho visto dagli applausi - evidenziando alcuni aspetti dell'impegno e della personalità del presidente Andreotti, che rischiano di perdersi nella mole degli auguri, del resto meritatissimi. Dire che Giulio Andreotti sia un testimone del tempo è davvero insufficiente e anche inutile. Andreotti è un "presente" del e nel tempo; nella sua vita non ha osservato come va il mondo in diversi momenti storici e politici, ma ha partecipato con sorprendente assiduità alle scelte che hanno determinato gli eventi; ha contribuito ad affrontare problemi nazionali con lo sforzo costante di superare le difficoltà e spesso anche le insufficienze di una società italiana non sempre pronta. Forse adesso, a novant'anni, è soprattutto un osservatore e tuttavia non si nega mai alla richiesta di un parere che sa offrire, rimanendo ancorato alla razionalità dei fatti. Nella traversata del grande mare dell'attività pubblica ha dovuto superare non poche difficoltà dovute ad avversioni personali perché, come accade in politica, i problemi in questo senso sono strutturali e - sono parte del mestiere. In realtà, nella vita politica risulta vero quello che talora Andreotti stesso ha ricordato, citando Cicerone di cui è un grande cultore, e che cioè la politica non crea le amicizie, ma capita spesso che guasti anche quelle che ci sono. È in Parlamento dall'inizio dei lavori del nostro più alto consesso democratico e la sua vita è una presenza, come già è stato ricordato prima da altri colleghi. Una personalità poliedrica, per molti misteriosa: politico, uomo di cultura, giornalista, uomo di fede. Ha vissuto ed osservato con interesse gli avvenimenti ed è diventata famosa la sua capacità dì prestare attenzione. Andreotti non è mai un distratto. Riconosce sempre l'obiettivo e non finge attenzione dove non c'è interesse a prestarla. Non c'è riunione alla quale Andreotti partecipi senza prendere appunti che, data la costanza del suo scrivere, sono puntigliosi e attenti ai dettagli, quei dettagli nei quali si insinuano elementi decisivi di conoscenza e di interpretazione delle diverse Ho sempre invidiato la sua capacità di registrare anche in poche righe le giornate sul suo diario. Questa caratteristica non è un vezzo e c'è stato un tempo in cui, lo so Presidente, la sua la sua preziosa agenda, ben annotata le è servita per difendere la sua dignità, il suo prestigio e la sua persona. Così, la statura del personaggio Andreotti non è legata alla sua età, ma alla sua competenza e assiduità nell'esercitare il ruolo che nel tempo gli è toccato. Certamente, anche l'età conta, perché una persona come lui ne ha viste proprio tante, come ormai pochissimi altri sulla scena politica. Andreotti ha percorso una strada da un certo punto di vista del tutto lineare. È passato dal movimento dell'Azione cattolica, nei suoi rami, per giungere a fianco di De Gasperi al centro della direzione politica del Paese negli anni della ricostruzione. Gli incarichi governativi, e soprattutto quello di Presidente del Consiglio, gli hanno fatto attraversare tutte le diverse fasi dei 60 anni della nostra democrazia, sempre con l'ancoraggio ai fondamenti della Costituzione. Le crisi delle alleanze, la guerra fredda, il terrorismo, le crisi economiche, ed infine il passaggio alla cosiddetta seconda Repubblica. Presidente, quante volte le è stato rimproverato cinismo e, a causa delle sue battute spesso fulminanti, un eccessivo distacco dalla realtà. Ma c'è voluto molto coraggio a fronteggiare certe realtà! Non so quanti colleghi in quest'Aula possono riconoscerle la forza della sua scelta quando con un Governo monocolore nel 1976, perché nessuno ci stava ad accolarsi quella grana, ha affrontato una crisi gravissima che ha richiesto di impegnare le riserve auree del nostro Paese per avere il prestito dalla Germania. Che esempio anche per la crisi di oggi! I diversi ruoli assunti dimostrano come il suo carattere di osservatore si sia fuso completamente con quello dell'attore, dimostrando che si può servire il Paese in diverse dimensioni; da posizioni istituzionali di prestigio, ma anche da umili e quotidiane attenzioni ai problemi della gente. Mi piacerebbe chiedere alle persone che il sabato e la domenica si recavano al suo studio un giudizio su Andreotti; persone umili, provenienti dalla campagna romana, povera gente proveniente dai quartieri più periferici e popolari della città. Durante la mia esperienza di Vice Sindaco di Roma il Presidente mi ha presentato spesso le esigenze più elementari della gente, soprattutto dei giovani, non certamente per un tornaconto personale o elettoralistico, bensì per l'ansia di garantire alcuni diritti fondamentali. Nonostante il crescente rilievo assunto nei diversi ruoli, non ha mai voluto assumere una carica importante di partito, limitandosi al più ad essere un *leader* di corrente, anche competitivo. Tra gli incarichi di governo, quello di Ministro degli esteri è diventato negli anni quasi più importante di tutti gli altri, importantissimi, rivestiti. Con la sua direzione degli affari esteri il nostro Paese è riuscito a mantenersi in una zona di confine dell'area politica occidentale, in una posizione di vera difesa della pace. La fedeltà alla Costituzione ha creato l'argine entro cui l'azione della politica italiana si è svolta senza oltranzismi. Andreotti è stato ed è ancora protagonista della politica internazionale perché ancora oggi molti Capi di Stato di passaggio a Roma fanno tappa da lui per confrontarsi con lui ed avere magari ancora consigli. Del resto, la sua assidua partecipazione ai lavori della Commissione esteri del Senato continua a testimoniare quanto, come De Gasperi, Andreotti sia convinto che dalla politica estera arrivino sostegno e fondazioni anche per gli interessi della politica interna. Da letterato, il Presidente partecipa alla Società dantesca, al Certamen ciceroniano ed ad altro ancora. Ha scritto moltissimo, è già stato ricordato; la sua è una cultura vissuta mai ostentata come valore astratto o di moda. Lo anima certamente il desiderio di voler trasmettere ed affidare alle generazioni future la testimonianza di stagioni politiche che, pure in mezzo a tante difficoltà, hanno costruito la nostra democrazia. Credo corrisponda a questo intento anche la sua decisione di consegnare, per mettere a disposizione di ricercatori e studiosi, il suo archivio personale all'Istituto Luigi Sturzo, prestigioso luogo storico, che conserva la memoria di molti politici cattolici che hanno segnato le vicende del nostro Paese. Sintetizza la sua *verve* giornalistica ed il suo impegno divulgativo con la direzione del mensile «30 Giorni» che ha come sottotitolo «Nella Chiesa e nel mondo» e che viene diffusa e tradotta in sette lingue. È una dimensione imprescindibile, essenziale nella sua vita, la testimonianza di fede cristiana vissuta quotidianamente e che, senza dubbio, ha sorretto la sua forza interiore quando ha dovuto affrontare le tremende vicende che l'hanno colpito negli ultimi anni. Ma è stato un politico esemplare nell'interpretare la laicità delle istituzioni e questo è un aspetto non abbastanza valorizzato. Basti ricordare che cosa ha rappresentato la firma della legge n. 194. Non c'è un'espressione che possa riassumere interamente il profilo, l'attività, la personalità di Andreotti. Anzi, Presidente, so che le mie parole sono state povere e insufficienti non solo a causa del poco tempo che abbiamo a disposizione. Mi pare di vederla sorridere anche sotto i baffi che non ha, dicendo che ci mancava solo «il coccodrillo da vivo». Ridiamo con lei, ridiamo delle sue battute, che sono uno degli aspetti che la rendono tanto simpatico agli italiani, anche quelli che hanno una valutazione politica diversa dalla sua, anche a quella gente di ogni ceto che sa che lei ha partecipato a regalarci questo grande Paese, che ha vissuto in pace ed è rispettato nell'arena di tutti i Paesi civili e democratici del mondo. Auguri, *ad multos annos* ancora, Presidente. Signor Presidente, a nome di tutto il Gruppo del Popolo della Libertà mi unisco

ha detto: «non mi piacciono le biografie da vivo, però capisco che ci si occupi della mia vita; in fondo, in un certo senso io sono postumo di me stesso». Una frase autoironica che segna la valutazione di una personalità - come è stato detto dal presidente Schifani e dai colleghi che mi hanno preceduto - ma anche la storia italiana. Voglio anch'io sottolineare alcuni aspetti da indicare alla pubblica opinione, ai cittadini, che vedono in Andreotti uno dei simboli della storia italiana

Mi dicono che fosse molto attento a valorizzare l'impegno dei singoli colleghi, a valutare i loro interventi, le loro presenze, prendendo nota in maniera diligente dei meriti e delle eventuali mancanze, ma soprattutto dei meriti di ciascuno.

in una delle tante interviste rilasciate in questi giorni di celebrazioni, il presidente Andreotti ha detto una cosa molto importante per l'attività parlamentare, che egli ama più le Commissioni

Come è stato ricordato, anche in questi giorni egli non ha fatto mancare la sua presenza, il suo consiglio e la sua opinione, come fa abitualmente. Credo che questo sia un esempio per tanti giovani parlamentari che spesso mostrano insofferenza o frustrazione per il quotidiano lavoro parlamentare, che invece è importante, prezioso e va vissuto con spirito di servizio come il presidente Andreotti, carico di gloria e di incarichi, potrebbe non fare e invece fa, essendo anche in questo esempio esempio per coloro che nel tempo sono entrati in Parlamento. Dell'uomo di Governo si è detto molto. Sono stati ricordati gli incarichi. È capitato a tutti di convenire sulle sue scelte o di non acconsentire ad esse. Saremmo ipocriti nel non ricordare che il presidente Andreotti, protagonista della lunga storia del dopoguerra, ha raccolto ampi consensi e ha spesso suscitato dissensi, come tutti i grandi personaggi.

fin dal suo incarico di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, un attivo movimentatore di idee, di personaggi, di situazioni, di istituzioni che oggi lo portano ad essere un ascoltato *opinion leader* in tanti campi della vita culturale e civile della Nazione: dai primi momenti del cinema italiano del dopoguerra ad Arcinazzo, ad incontri che cercavano di ricomporre una lacerata vita italiana che aveva bisogno di ritrovare momenti di coesione dopo guerre civili e scontri drammatici. Voglio del giornalismo, l'uomo dei libri, lo scrittore che ha regalato riflessioni importanti ma anche analisi spesso ironiche ed autoironiche, anche della vita parlamentare, dei suoi aspetti più pungenti, riflessioni tra le più serie ed importanti, espresse sempre con una grande autoironia. Il presidente Andreotti tempo fa disse: «Mi hanno attribuito praticamente tutto, tranne che le guerre puniche». Chissà che nella lunga vita che lo attende ancora qualcuno non gli attribuisca qualche responsabilità anche in questa materia.

ha atteso con pazienza e forse troppo a lungo - lasciatemelo dire - che i giudizi dessero ragione alla sua perseveranza.

nel quale confluiscono tante esperienze, tante culture, tante sensibilità, alcune più vicine, altre meno alla lunga esperienza politica del presidente Andreotti, ma tutte rispettose della sua persona

come concittadino, come abitante dello stesso quartiere e frequentatore della stessa parrocchia, come compagno di scuola ma, ovviamente, soprattutto, come Presidente del Gruppo che ho l'onore di presiedere, le rivolgo ancora una volta tanti auguri, presidente Andreotti.

pensare di percorrere la storia della prima metà del secolo scorso, quando il giovane Andreotti si turbava a vedere i turbamenti di un Papa, prima ancora di Pio XII, che assisteva personalmente. la storia della guerra e quella del dopoguerra. Una presenza costante, per me che sono nato nel 1950, di una persona che già era ai vertici dello Stato e che rappresentava - lo dice lui stesso - la presenza fisica con altri personaggi: Vittorio Emanuele Orlando, Nitti. Andreotti scrive di di fronte a questi padri della Patria, protagonisti della prima guerra mondiale, della storia d'Italia, intimorito a sedere in Parlamento con questi monumenti della storia del nostro Paese. Era l'Italia che usciva dalla guerra; era l'Italia dei personaggi come De Gasperi, di cui Andreotti fu uno strettissimo collaboratore; era l'Italia a cui tantissimi di noi guardavano. Io mi sono iscritto nel 1968 alla Democrazia Cristiana - non ne faccio mistero avevo in mente il presidente del Consiglio De Gasperi, il presidente del Consiglio Pella, il presidente del Consiglio Scelba, tutta la storia degli anni '50 e '60, la storia democratica di uomini che avevano saputo nel contempo essere rigorosamente antifascisti, ma anche molto fermi nei confronti del comunismo di allora, e che avevano tracciato una strada di democrazia per il nostro Paese. Credo che nei vari interventi dell'Andreotti politico, statista, Ministro, Presidente del consiglio, scrittore, cultore di scienze umane sia stato detto tutto; vorrei solo sottolineare un tratto che poi nelle persone è l'aspetto più importante. Quando recentemente - lo avrete letto tutti - è iniziata una campagna diffamatoria e vergognosa nei confronti del Senato, del comportamento dei senatori che magari quando votano fanno anche qualcos'altro, mi è venuto da pensare che Andreotti l'ha sempre fatto; partecipare, intervenire, votare, scrivere, lavorare, perché chiunque si è rivolto a lui e gli ha scritto qualcosa ha ricevuto di suo pugno una risposta. Ciò denota un grande rispetto per la gente, un grande rispetto per il rapporto con chiunque, possa essere il Sommo Pontefice - ed è stato ricordato - o l'ultimo degli elettori, non quando aveva bisogno delle preferenze. Come senatore a vita non ne ha bisogno, ma la passione politica continua a portarlo a coltivare questo rapporto con la gente per risolvere i problemi delle persone. A Giulio Andreotti faccio un augurio in una nicchia particolarissima che non è stata ancora ricordata, che ci sia la possibilità di trovare quelle due buste mancanti di storia postale del 1870. Andreotti, grande cultore di storia postale, ha tutti i giorni di quell'anno fatidico, il 1870, di buste che partirono in quell'anno da quando lo Stato della Chiesa diventava Stato italiano. Quindi, gli auguro di poter continuare a coltivare le sue passioni. Faccio verificare a tutti un fenomeno che capita raramente in Parlamento. È vero, è difficilissimo attirare l'attenzione dei colleghi. Tutti noi invece sappiamo una cosa importante e significativa, ossia che quando Giulio Andreotti si alza in piedi, quando parla, quando parla, l'Assemblea lo ascolta in religioso silenzio, perché tutti sappiamo che quando interviene abbiamo sempre qualcosa da imparare dalla sua esperienza e dalla sua limpida storia democratica. Allora, lunga vita al senatore Andreotti, che rimanga ancora fra di noi per darci il frutto della sua esperienza e della sua capacità.

Presidente, non voglio davvero abusare del tempo delSenato, ma non posso non ringraziare per quello che ho udito. Potrei - conoscendomi meglio di quanto mi conoscete voi - fare tutto un controcanto, riferendo tutta una serie di difetti e di mancate occasioni positive che

aperture di altro genere, ne sono stato però sempre progressivamente attratto. Se ho un rammarico è quello di non aver contribuito abbastanza a fare quello che manca, cioè far conoscere meglio l'attività reale dei due rami del Parlamento all'opinione pubblica, che è distratta. Infatti, se un giorno

il resto, prima ho ascoltato con una certa esitazione, perché ho assistito a molte commemorazioni, ma quelle da vivo sono un po' diverse!

assolutamente in armonia con la propria coscienza. Credo che il concetto che qualche volta polemicamente - ma non è una cosa nuova, è sempre stato così - si ha della vita pubblica, considerata quasi in un modo negativo, in un modo più critico

di rasserenamento graduale, ma costante, con un indirizzo molto preciso, questo lo si deve molto al lavoro silenzioso, ma estremamente positivo, che viene fatto dal Parlamento. Ringrazio Dio di esserne partecipe da tanto tempo.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12,

Avevo pregato i colleghi di stare seduti al proprio posto. Ve lo chiedo per cortesia.

proponiamo di sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 13. Riteniamo infatti che la norma sia vaga e indeterminata, come invece non deve essere una norma penale. Prevedere un aumento di pena per i fatti commessi nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori significa

Non si capisce poi l'aggravante che viene introdotta dal comma 3 per il delitto di violenza sessuale se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze della scuola frequentata dalla persona offesa.

della comune abitazione da parte del soggetto e della vittima,

che è molto diffusa, su cui purtroppo vi è una zona d'ombra nel nostro sistema. Mi riferisco al reato di adescamento di minorenni attraverso la utilizzazione della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

i minori esposti a questa particolare insidia che viene loro portata attraverso la rete Internet.

in atto nel territorio campano, in particolare nella provincia di Caserta, che rappresenta non un punto di arrivo, ma comunque una tappa importante. ha avuto modo di chiamare personalmente il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Siazzu, per manifestargli, a nome proprio e dell'intera Assemblea, il compiacimento per la prodigiosa estrategica operazione di cattura realizzata dall'Arma.

È scritto anche nella Costituzione che il domicilio è inviolabile e pertanto la propria abitazione non può essere assoggettata a furti, aggressioni, rapine e ad ogni tipo di violazione di domicilio. Per questo motivo siamo intervenuti su questo reato di violazione di domicilio introducendo un minimo edittale di sei mesi (prima non era previsto un minimo edittale) e introducendo l'arresto obbligatorio in flagranza per le ipotesi di furto con travisamento e con armi (anche se non usate), ipotesi di furto che sono tipiche nelle nostre abitazioni.

parla di pene diminuite per chi si adopera concretamente affinché il minore riacquisti la propria libertà oppure si adopera perché l'attività delittuosa non venga portata ad ulteriori conseguenze e nei casi di aiuto all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria; e nella parte finale si segnala che la pena viene diminuita anche per i casi in cui si eviti la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore. Ci sembrerebbe idoneo introdurre un allargamento nel senso che, nei casi di ravvedimento e quindi di concreto aiuto da parte della persona alla polizia o alla magistratura per impedire sequestri di qualsiasi persona, che sia minore o non, credo sarebbe un risultato positivo e che anche da parte del Governo e della maggioranza non dovrebbe esserci nulla in contrario. Riguarda - lo ripeto - l'aiuto per evitare sequestri di persona, sia minorenne che maggiorenne.

cercherò di rubare poco tempo all'Assemblea, ma ho la necessità di illustrare con un po' di precisione questo emendamento che si propone, introducendo una norma attuativa alla legge 18 aprile 1975, n. 110, che unitamente al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, disciplina il controllo delle armi e delle munizioni, di regolamentare in modo chiaro e trasparente la vendita e l'uso dei dispositivi di autodifesa di *oleoresin capsicum* nei cui riguardi il Ministero dell'interno si è già espresso, definendolo infatti privo di «attitudine a recare offesa alla persona». I problemi relativi alla legittimità di tali strumenti sono, infatti, determinati dalla complessità della legge n. 110 del 1975 e dalla confusione generata dalle sue successive modifiche e integrazioni, succedutesi nel tempo, nonché dalle decine di circolari interpretative emanate dal Ministero dell'interno. In realtà, il Ministero dell'interno ha già autorizzato la libera commercializzazione di due prodotti contenenti il principio in questione, in quanto non classificabili armi comuni, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 110 del 1975, tale autorizzazione è stata rilasciata con una circolare del 9 gennaio 1998 e con la comunicazione del 25 giugno 1998, del Dipartimento della pubblica sicurezza-direzione centrale degli affari generali-divisione armi ed esplosivi, condividendo il parere positivo espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge n. Va messo in evidenza che tale commissione è l'unico soggetto qualificato per esprimere una valutazione sulle caratteristiche delle armi e sulla loro attitudine a recare offesa alla persona. La confusione riguardo la legittimità della vendita e del porto degli spray per autodifesa nasce negli anni Novanta, quando in Italia, ma soprattutto in Europa, vengono vengono immesse sul mercato due tipologie di prodotti: gli spray contenenti aggressivi chimici, comunemente conosciuti come "CS", con effetti lacrimogeni, utilizzati dalle forze di polizia;

In realtà, lo spray contenente "CS", cioè quello molto diffuso in Europa, poiché contenente un aggressivo chimico è sempre stato considerato assolutamente illegale in Italia

tale prodotto viene liberamente venduto negli altri paesi dell'Unione europea, persino nelle tabaccherie, e sarebbe comunque, a prescindere dalla normativa italiana, di facile reperibilità per i soggetti malintenzionati. Purtroppo, molti organi di polizia, confondendo i due prodotti, hanno avviato procedimenti anche nei confronti di soggetti che commercializzano e portano il prodotto contenente il principio dell'*oleoresin capsicum* che, invece, essendo un prodotto organico, non è classificabile come aggressivo chimico e come tale è stato valutato positivamente dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa e penale ha sancito la differenza tra le due sostanze, emettendo sentenze di assoluzione nel caso specifico dell'*oleoresin capsicum*. È comunque evidente che per l'ordinamento penale italiano un uso dello spray finalizzato a commettere reati comporterebbe la sua considerazione come arma impropria, con tutte le conseguenze già previste dalla legge, come per qualsiasi altro oggetto che venisse utilizzato come strumento di aggressione. L'intervento normativo si rende quindi necessario affinché sia emanato dal Ministero dell'interno uno specifico regolamento, ispirato a criteri di trasparenza, per l'immissione sul mercato di dispositivi di autodifesa che nebulizzano il principio attivo naturale a base di *oleoresin capsicum* e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona, sulla base di quanto già valutato come idoneo

di attuazione che integra quanto previsto dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come prima sostituito dall'articolo 1 della legge n. 36 del 21 febbraio 1990. E fin qui la parte tecnica, signor Presidente. Ma non sfugge a nessuno che la preoccupante crescita di fenomeni di violenza, in special modo contro le donne, e l'agghiacciante lista di morti annunciate o di violenze che esplodono imprevedibili pongono alla nostra attenzione cosa fare, tra le tante cose da fare, nell'ambito di una migliore organizzazione della sicurezza del nostro Paese, anche da parte nostra. Sappiamo bene che, nonostante gli sforzi di questo Governo e le risorse messe in campo, non ci può essere un poliziotto in ogni angolo di strada. Ha fatto bene a ricordarlo il senatore Bianco, quando, qualche giorno fa, in una dichiarazione, a proposito dell'esame di questo provvedimento, ha ricordato

anche da questo punto di vista, che dobbiamo poter fare le nostra parte, puntando ad una migliore normativa. E ringrazio il Governo per aver voluto ascoltare le ragioni che tante donne e associazioni femminili

di difesa personale, però, ciascuno di noi - in modo particolare, le donne italiane - potrà girare per le strade sapendo di essere al sicuro da un'emergenza, in

consentiti il porto e la vendita di bombolette spray per autodifesa e vi è un conflitto giurisprudenziale nell'applicazione delle normative che

migliore e una parte della giurisprudenza ne hanno invocato una rideterminazione sul piano della tassatività della norma penale.

dei rapporti giuridici e, in particolare, la tassatività delle norme penali incriminatrici, evidentemente oggetto di una tutela sottolineata da parte della Costituzione della Repubblica.

- se mi si passa il termine - giuridicamente e politicamente più ipocrita, ma sotto il profilo politico e dell'impatto è parimenti grave. Infatti, signor Presidente,

ma quando trattiamo un tema così delicato e complesso come quello dell'immigrazione dobbiamo anche avere l'accortezza, nel momento in cui interveniamo profondamente sotto il profilo delle norme penali e sanzionatorie, di capire quale impatto queste abbiano e se siano oggettivamente utili e funzionali a contrastare il problema. Nel caso che ci riguarda, ci troviamo di fronte all'ipotesi di

e quindi del mantenimento della presenza fisica dell'extracomunitario all'interno del territorio dello Stato. È noto a tutti il principio di irretroattività della norma penale, per cui la prima questione è come si possa accertare se l'ipotesi dell'ingresso o della permanenza illegale nel territorio dello Stato sia cronologicamente anteriore o successiva all'entrata in vigore della nuova norma incriminatoria.

sostenuto questa posizione e non la smentisco oggi per ragioni di coerenza. Ma, proprio invocando quel principio in forza del quale non vi è la possibilità di un accertamento reale della condizione per la quale scatta la sanzione penale,

e la permanenza nel territorio dello Stato sia antecedente o meno all'entrata in vigore della norma. Poiché questa norma, correttamente, non si applica alla condizione diversa, cioè al respingimento alla frontiera,

perché il comma 4 della nuova versione dell'articolo 19 prevede che ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero, denunciato ai sensi del comma 1, non è richiesto il nulla osta dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3 dell'articolo 13 del testo unico della legge sull'immigrazione

si procede all'espulsione del clandestino. Tradotto in termini molto semplici questo significa che la norma è ipocrita e più pericolosa di quella precedente, perché consente l'espulsione anche di soggetti la cui condizione di irregolarità è controversa

senza ottenere alcun risultato se non quello di aumentare il livello del contenzioso intasando gli uffici giudiziari, di rendere ancora più difficile il compito delle forze dell'ordine rispetto a questo tema

in violazione assoluta dei principi e delle norme costituzionali di uguaglianza, ma sia soprattutto inutile perché aggrava il procedimento, introduce una norma ipocrita ed odiosa che non serve a contrastare l'immigrazione clandestina ma solo a mettere l'ennesima bandierina populista e demagogica su un tema che invece è epocale, drammatico e necessita di interventi diversi. La norma, pertanto, non ci può trovare consenzienti, perché credo che questo non sia un modo serio, decoroso e dignitoso

contiene un riferimento a norme che non esistono nel nostro ordinamento. Infatti il comma 3 fa riferimento alla procedura che si applica ai processi penali; si richiamano gli articoli 20-*bis*,

non esistono. La Commissione quindi ha approvato una norma facendo riferimento ad articoli che non esistono. Il Governo, che se ne è accorto dopo che sui giornali l'ex procuratore aggiunto di Torino, Bruno Tinti, aveva ironizzato su questo infortunio, ha presentato un emendamento

sappiamo che il disegno di legge originario prevedeva il reato d'ingresso illegale nel territorio dello Stato, sanzionandolo con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

la sanzione, prevedendosi non più la reclusione da sei mesi a quattro anni bensì un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

sostiene che il processo per 49.050 ingressi illegali costa 650 euro per il gratuito patrocinio,

che la platea dei processandi non è più di 49.000 persone con un costo di 31 milioni di euro, bensì di 600.000 o 700.000 persone tra

Sapete cosa significa fare 700.000 processi pagando un costo stimato dal Governo in 650 euro a processo? Significa che ci stiamo accollando un costo di 400 milioni di euro per fare dei processi totalmente inutili. Applicandosi la normativa e quindi le disposizioni e le sanzioni che può adottare il giudice di pace, poiché la sanzione sanzione dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro è francamente impensabile (è soltanto risibile pensare che colui che faccia ingresso illegalmente in Italia paghi l'ammenda di 10.000 euro per farsi espellere), questa sanzione chiaramente non potrà essere applicata. Cosa potrà fare a quel punto il giudice di pace? La legge stabilisce che qualora l'ammenda non possa essere applicata o comunque non venga pagata, il giudice di pace deve convertire questa pena. In cosa può convertirla? In lavoro socialmente utile. L'irregolare però non può svolgere un lavoro socialmente utile perché non ha neanche una posizione assicurativa Allora cosa prevede la legge? Che qualora non si paghi l'ammenda e non si possa fare la conversione nel lavoro socialmente utile,

ossia l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione nei giorni di sabato e domenica. Ma voi riuscite ad immaginare l'irregolare che viene condannato a rimanere nella propria abitazione nei giorni di sabato e domenica! Stiamo facendo tutto questo, spendendo 400 milioni, per fare questo ridicolo Colui che sbarca senza dimora lo processiamo e lo condanniamo a rimanere in una dimora, che non ha, nei giorni di sabato e domenica, perché gli altri giorni è libero! Questo può fare il giudice di pace. di pace. A cosa serve? Non esiste più l'espulsione amministrativa? Non si applica agli irregolari che soggiornano nel nostro Paese l'espulsione amministrativa? Non è stato detto anche recentemente dal ministro Maroni che coloro che stavano sbarcando a Lampedusa sarebbero stati subito rimpatriati? Allora si può fare? Per quale motivo dobbiamo fare questo ridicolo processo, con questi enormi costi, per arrivare al risultato dell'espulsione che posso già oggi applicare attraverso la norma che già esiste. Ecco perché riteniamo

insistiamo e sollecitiamo, signor Presidente, attraverso i suoi poteri, anche la Commissione bilancio a non fidarsi dei numeri

delitto così grave per cui era previsto il giudizio direttissimo. Si sarebbero dovuti processare circa 50.000 ingressi abusivi, per cui la magistratura sarebbe stata bloccata con i processi per direttissima esclusivamente su questo reato.

sicurezze per i cittadini, quali la criminalità diffusa e la criminalità organizzata, c'era dell'altro. Per la verità mi ero anche compiaciuto sotto questo profilo quando poi si è cominciato a parlare di eliminare Non so se mi devo compiacere con le osservazioni che furono fatte in sede di Commissione in quella occasione, perché non c'erano solo i processi da compiere, ma ci sarebbero state anche le carceri da costruire

posizione, anche facendo tesoro delle mie precedenti esperienze e di quello che era stato detto dal Capo dell'ufficio immigrazione americano, secondo il quale non era questo il modo di combattere l'immigrazione clandestina.

mandato i nostri uomini e le nostre navi per impedire la partenza dei migranti. Così si sarebbe dovuto fare anche in questo caso: gli sbarchi clandestini che ci sono stati a Lampedusa

che quando l'immigrato arriva in Italia gli si debba chiedere per prima cosa se ha la carta di credito per pagare l'eventuale contravvenzione a cui verrà condannato. Ci troviamo quindi di fronte a uno di quei reati assolutamente inutili sotto ogni profilo.

perché stabilire un reato quando ciò non accade neanche negli Stati Uniti d'America, che è la Nazione che ha fatto maggiori esperienze sull'immigrazione clandestina? Ricordo che quando uno dei miei colleghi chiese al Capo dell'Ufficio immigrazione

usare le somme che sono state stanziate per bloccare l'immigrazione clandestina, per stabilire convenzioni internazionali con i Paesi da cui queste persone migrano e per aiutarle a rimanere nei luoghi da cui provengono.

rendere conto che più si appesantisce la magistratura con questi reati, meno sarà efficiente la giustizia. Noi siamo meno efficienti degli altri perché abbiamo un numero di reati spropositato e un numero di reati di qualità veramente

l'opportunità di sottoscrivere questo emendamento che introduce il reato di tortura. Mi auguro che, oltre ad ascoltarmi, il sottosegretario Mantovano

ma potrebbe essere, quantomeno, l'occasione per introdurre un reato che l'Italia aspetta da oltre vent'anni, cioè da quando abbiamo sottoscritto la Convenzione internazionale contro la tortura. L'emendamento 34.0.100 per il momento ha già una trentina di sottoscrittori

si è più volte appellata direttamente al Presidente del Consiglio, quello stesso presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che nel 1994 si appellò perché in Italia fosse introdotto il reato di tortura. Allora, perché non cogliere l'occasione di questo disegno di legge e di questo emendamento, che con generosità vi abbiamo proposto e sul quale chiediamo al Governo di esprimere un parere positivo o, quantomeno, di rimettersi all'Aula nel rispetto di un Parlamento che potrebbe colmare quel vuoto legislativo

dell'Italia, in cui si definisce tortura ogni atto mediante il quale siano inflitti intenzionalmente ad una persona dolori o sofferenze gravi, sia fisici che mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso

a condizione che la sofferenza o il dolore siano inflitti da o su istigazione o con il consenso o l'acquiescenza di un pubblico ufficiale o altra persona che svolga una funzione ufficiale.

io termino qui e so che, in parte, posso essere andata fuori dall'ambito di competenza degli emendamenti all'articolo 19, però, visto che parliamo anche di come trattare gli immigrati, di come sanzionarli, di come punirli e di come mandarli ipoteticamente anche nelle nostre carceri, che sono in una situazione di degrado e di sovraffollamento, inviterei a fare attenzione ad introdurre nuovi reati ma ad introdurre, casomai, quelli che servono o che servirebbero anche all'Italia.

a fronte di una disposizione, quella di cui si sono occupati finora i colleghi con ricchezza di argomenti, che francamente che francamente suscita - volendo utilizzare un'espressione eufemistica - una straordinaria perplessità. Signor Presidente, la norma precedente, anch'essa già citata più volte e che prevedeva l'ingresso abusivo nel territorio dello Stato come un delitto, era norma, a nostro modo di vedere, esecrabile ma munita di senso. Con il disposto penalistico e processual-penalistico, infatti, costruito intorno alla fattispecie, la prospettiva che potesse trattarsi di una sorta di presidio dissuasivo al fine di ridurre l'impatto delle entrate illegali nel nostro territorio sembrava una tesi astrattamente sostenibile (dal nostro punto di vista assolutamente priva di qualsiasi prospettiva pratica per una serie di ragioni su cui non tornerò per non appesantire inutilmente l'intervento) nel quadro di una dialettica tra posizioni molto diverse. Ciò che è accaduto nel corso della storia parlamentare di questa norma lascia francamente lo dico con molta serenità - esterrefatti quanto allo strumentario tecnico-giuridico che assiste questo tipo di interventi. È stato già detto - ma voglio ripeterlo, evidenziando qualche altro piccolo dettaglio si tratta di una contravvenzione, punita con una pena pecuniaria ridicola, se si ha riferimento ai destinatari della norma, cioè soggetti nella stragrande maggioranza dei casi nullatenenti. Si tratta di una norma, gioiello di dottrina penalistica, non oblabile. Chiunque abbia dimestichezza con il processo penale e con le sue fumisterie sa che le contravvenzioni sono normalmente, salvo casi eccezionali, oblabili perché ciò risponde, in presenza di condotte ritenute comunque devianti, all'esigenza di accelerare il funzionamento della macchina processuale. In questo caso abbiamo una norma che, come bene ha detto il senatore D'Alia, qualificandola ipocrita e odiosa, caricherà in modo clamoroso gli uffici giudiziari. E questo tema è stato riccamente illustrato anche

si occupa - da una a due ore di lavoro, che potrebbero essere utilizzate presidiando il territorio, intervenendo nei confronti dell'autentica devianza sociale, anche quella posta in essere dagli immigrati - che esistono, nessuno lo nega, e a quelli dovremmo dedicarci - che commettono reati. Avremo invece forze di polizia - il sottosegretario Mantovano lo sa molto bene poiché egli stesso è all'interno della

Avremo uffici di polizia nei quali ci sono funzionari e sottufficiali abitualmente dediti al lavoro ed alla produttività (la maggioranza)

qualche funzionario non particolarmente incline all'attività investigativa o all'autentica repressione dei fenomeni di devianza troverà un facile rifugio statistico nella redazione di decine e decine di queste ridicole informative, per questo ridicolo e inutile che rimane in questa legge soltanto come emblema di un preconcetto ideologico, con una prospettiva vagamente e forse non troppo vagamente discriminatoria, e di cui francamente non sentivamo il bisogno.

vogliamo sottolineare la valenza di un'attività di questo tipo, specialmente in riferimento ad alcune Regioni e ad alcuni territori dell'Italia meridionale, a rischio notevolissimo proprio per quanto riguarda l'aspetto dell'immigrazione e dell'integrazione.

tipicamente mafiosa. L'emendamento 19.110 si rivolge quindi proprio ad un'attività di prevenzione generale e vuole sollecitare una collaborazione con i servizi di polizia giudiziaria e con le autorità giudiziarie di quei territori, per evitare effetti e conseguenze ancora più gravi. *(Applausi

dell'originale testo del Governo: si tratta, cioè, di far fare alle forze di polizia l'attività loro propria e non quella di ufficiali giudiziari.

fare i nomi degli assenti, posso certificare che il senatore Caligiuri da due ore non è in Aula eppure continua a votare. Se vuole controllare i tabulati, sicuramente scoprirà che è stato votato più volte per il senatore Caligiuri.

Faremo una verifica in occasione di queste votazioni e se il senatore Caligiuri, che non vedo, tra l'altro, dovesse risultare presente ripeteremo la votazione.

Il Senato è in numero legale.

fondamentale nel sistema di lotta all'immigrazione clandestina e illegale. Finalmente compiamo un passaggio importantissimo anche dal punto di vista culturale. Come sapete, colleghi, un *dossier* dell'Ufficio Studi del Senato, pochi mesi fa, ci ha fatto scoprire che Francia, Germania e Inghilterra considerano già l'immigrazione clandestina un reato e lo perseguono in maniera molto più pesante di quello che ci ci accingiamo a fare noi. L'unico Paese che non ha una fattispecie di rilievo penale è la Spagna che considera, però, l'immigrazione clandestina una violazione amministrativa gravissima, punita con una sanzione pecuniaria ben superiore a quella che noi introduciamo sotto forma di ammenda senza oblazione. Quindi, non si tratta di una norma razzista o antidemocratica o di una norma manifesto, come ho sentito dire, bensì di una norma fondamentale per porsi in linea con gli altri Paesi europei nella lotta all'immigrazione clandestina se la si vuole fare davvero, e noi intendiamo farla davvero.

cardine nella lotta all'immigrazione clandestina. Benissimo, partiamo da qui: innanzitutto occorre finirla con la storiella che

Il Partito Democratico crede che l'immigrazione debba essere regolare, e debba avvenire secondo i principi della legge, questa è la premessa.

tra il mezzo milione e un milione di immigrati che lavorano regolarmente nel nostro Paese, quasi senza eccezione, che sono in posizione di irregolarità. Dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza - l'onorevole Mantovano del resto è del mestiere perché è stato per cinque anni, e lo è di nuovo, in un posto cruciale al Ministero dell'interno - e riconoscere che è la stessa legge Bossi-Fini e i suoi meccanismi che determinano l'alto livello di irregolarità nel nostro Paese. i modi di ammissione legale nel nostro Paese non consentono l'incontro tra offerta e domanda di manodopera e quindi è vantaggioso per tutti, a cominciare dai datori di lavoro, che un immigrato arrivi regolarmente ma che permanga irregolarmente nel nostro territorio. Se non si riconosce questo, continueremo ad inasprire le sanzioni contro l'irregolarità, ma nello stesso tempo a non chiudere il rubinetto dell'irregolarità. Voglio

che prevedeva una condanna penale con la reclusione per coloro che si macchiavano di questo gravissimo reato; marcia indietro assolutamente clamorosa dovuta al fatto che la norma era inapplicabile inapplicabile e che quasi tutti i centri di opinione che contano in questo Paese (gli imprenditori, l'opinione pubblica,

quando si accerta una irregolarità e prima di procedere all'espulsione si debbono esperire vari tentativi. all'immigrato irregolare che non sia un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico - per inciso, mi domando quante centinaia di migliaia di badanti o di

deve essere concesso un periodo compreso tra i 7 e i 30 giorni per ottemperare volontariamente all'ordine di rimpatrio. Quindi, non espulsione di massa, che è inattuabile e che l'Unione europea non ci permetterebbe di fare,

Mi sembrerebbe più che naturale che ciò avvenisse. Invece il nostro Governo propone il pugno duro contro la stragrande maggioranza dei nostri irregolari.

prevede che durante il periodo di tregua si possa pretendere una garanzia finanziaria prima che l'espulsione venga eseguita.

fa molti più danni dei vantaggi che pensa di poter arrecare alla nostra società. Gran parte degli irregolari presenti nel nostro territorio sono persone in regola con la propria coscienza, nei rapporti sociali e nelle loro famiglie, l'idea che tutti debbano essere soggetti ad espulsione è davvero peregrina. Spero che questo Senato abbia un sussulto. Spero, ma non ci credo. per affrontare l'irregolarità il Governo debba tirare fuori altre armi diverse da quella dell'inasprimento delle pene e spero che prima o poi questa idea saggia si faccia strada.

al prolungamento fino a 18 mesi della permanenza temporanea nei centri. Ricordo a me stesso che, se non sbaglio, analogo trattamento in termini di custodia cautelare non si riserva né ai criminali comuni si associa ancora alla fideiussione bancaria e/o assicurativa per l'esercizio di un'attività imprenditoriale e alla omologazione, sotto il profilo del trattamento, dei cittadini comunitari stranieri agli extracomunitari. Qual è allora la questione, cari colleghi moderati del Popolo della Libertà? Voi state pagando un prezzo politico alla Lega, legittimo - onore al merito della Lega - ma che è lontano mille miglia dalla nostra posizione politica e credo anche da quella della stragrande maggioranza dei cittadini di buon senso che non la pensano come la Lega, che ha altri elettori di buon senso (per carità, non è un giudizio sulle persone). È però chiaro ed evidente che voi state assecondando l'introduzione di una norma odiosa, ipocrita ed inutile. Odiosa perché è un modo clandestino, questo sì, di reintrodurre, in violazione delle sentenze della Corte costituzionale, il principio e l'esecuzione immediata dell'espulsione per la sola denuncia, senza alcun accertamento giudiziario, della condizione di illiceità della permanenza nel territorio dello Stato, illiceità che, per quanto riguarda i fatti antecedenti all'entrata in vigore della norma, non è dimostrabile. State dicendo che State dicendo che tutto ciò lo può fare, con tutto il rispetto, il giudice di pace. State dicendo che intanto il clandestino, sia regolare che irregolare, se ne va, poi se ne parlerà.

nella disciplina dell'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro extracomunitario determina contenzioso sull'accertamento della titolarità e della legittimità della permanenza all'interno del territorio dello Stato.

pur avendo costi elevati ma una certezza sui tempi di esame e di rilascio, prevedeva l'introduzione di un costo aggiuntivo, così come ipotizzato sempre in via sperimentale per la carta d'identità elettronica. Ma cosa c'entra tutto questo con la condizione di regolarità dell'extracomunitario? Allora, quando per un fatto culturale asseverate questo tipo di scelte, non fate altro che prestare il fianco a quella polemica che non fa solo la Chiesa legittimamente, ma che fanno che non fa solo la Chiesa legittimamente, ma che fanno tutte le persone di buon senso che sostengono che bisogna distinguere l'immigrazione legale e regolare da quella irregolare. Questo non è un modo per distinguerla; questo è un modo ed un approccio culturale che assimila, che omologa fattispecie diverse e che quindi fa di tutta l'erba un fascio e non aiuta a risolvere i problemi del contrasto all'immigrazione clandestina. Queste sono le ragioni politiche per le quali votiamo contro l'articolo 19 e spero che qualche senatore del Gruppo

è piuttosto pittoresco il contesto di questo dibattito dal momento che si sostiene in quest'Aula la possibile esistenza dell'ipotesi per cui i cittadini italiani dovrebbero rispettare le norme giuridiche dello Stato di diritto e questo stesso obbligo non dovrebbe essere ascritto ai cittadini extracomunitari che entrano nel nostro Paese. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale hanno il dovere di conformarsi alle leggi vigenti del nostro Paese secondo il principio antico dello Stato di diritto, sia che questo si coniughi nell'espressione tedesca del *Rechtsstaat* o dello Stato di diritto francese o italiano, l'*État de droit*, o dello Stato di diritto inglese, *the Rule of law*. Voglio anche aggiungere che una recente legge approvata nel Regno Unito, la *Human rights act*, concede a quel Paese la possibilità di intervenire su questa materia con dei limiti che sicuramente non sarebbero compatibili con i princìpi della nostra Costituzione, in particolare con l'articolo 13. Allora, il dilemma che dovremmo sciogliere in quest'Aula è il seguente: capovolgere tutti i postulati dei più antichi padri del diritto moderno dello Stato di diritto, a cominciare da Hans Kelsen, cioè dovremmo sostenere la tesi che, di fronte ad un precetto che impone agli stranieri stranieri di regolarizzare il permesso di soggiorno nel nostro Paese e di renderlo entro otto giorni, poi in violazione di questo presupposto non ci dovrebbe essere una sanzione. Noi reintroduciamo, a seguito di un precetto, una sanzione che è perfettamente coerente con l'ordinamento giuridico del nostro Paese. Non abbiamo cambiato idea sull'illecito coerentemente, con la sistematica del codice Rocco del 1931, abbiamo applicato una sanzione di natura contravvenzionale alla violazione di obblighi amministrativi. Questa è la ragione giuridica che è conforme al principio di ragionevolezza delle leggi, per cui abbiamo introdotto l'ipotesi contravvenzionale. D'altra parte, la norma che introduciamo era già prevista nell'articolo 142 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, quindi trova conferma, ragionevolezza e sopratutto coerenza con il sistema giuridico del nostro Paese, ma in particolare con le sentenze della Corte costituzionale

che è un obbligo etico e morale, ma soprattutto civile, in primo luogo rispettare le leggi dell'ordinamento di un Paese civile e avanzato come l'Italia e poi richiedere quelle misure di solidarietà che all'interno di queste leggi approviamo. *(Applausi dal Gruppo affrontiamo questo problema perché nei due anni precedenti a questa legislatura, nel 2006 e nel 2007, sono entrati illegalmente in Italia 600.000 cittadini stranieri e c'è un problema serio di ordine pubblico e soprattutto di garanzia dei livelli di sicurezza del nostro Paese. Noi non abbiamo compresso i compresso i diritti fondamentali di libertà, che invece tentiamo di garantire, perché evidentemente esiste un *prius* rispetto a queste misure, che è la necessità di garantire i diritti fondamentali dei cittadini di questo Paese. Poco fa il senatore Mazzatorta, parlando della misura relativa alla tutela e alla protezione del domicilio, diceva che quella misura si riferisce alla protezione fisica del domicilio. Non è così: il domicilio e la libertà personale sono espressione di tutela della libertà e della dignità delle persone. Noi attraverso queste misure garantiamo questo diritto fondamentale, che è di tutti i cittadini e che, soprattutto, si radica nella storia costituzionale d'Europa d'Europa e nelle politiche che in Europa fa uno dei più grandi partiti, che è il Partito Popolare Europeo, al quale il nostro partito è iscritto. La nostra è una politica europea, è una politica di libertà, è una politica di civiltà. *(Applausi

La situazione oggi, con riguardo agli stranieri che entrano nel nostro Paese illegalmente, è disciplinata da una legge, la

11 parla di straniero «che è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera» e di straniero «che si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto». Quindi c'è lo strumento per intervenire. Voi oggi parlate in termini di rivoluzione culturale e dite che no, deve essere reato.

Noi immettiamo nel nostro sistema centinaia di migliaia di processi che riguarderanno le badanti. Questa norma si applicherà infatti proprio a quelle persone che versano in una situazione di irregolarità e che verranno processate perché nel nostro Paese l'azione penale è obbligatoria; non sarà nemmeno discrezionale: dovranno essere ricercate e processate. E coloro che daranno loro lavoro

dell'irregolare dandogli lavoro. Sicché noi faremo centinaia di migliaia di processi a carico di persone che versano in situazione irregolare e dei loro datori di lavoro: centinaia di migliaia di persone. Penso che qualcuno ci sarà anche in quest'Aula. Cominciasse subito a preoccuparsi, perché il reato a lui ascrivibile

Questa è la conseguenza. Ci saranno centinaia di migliaia di processi per il nulla, altro che bandiere, altro che principi e svolta culturale! State facendo qualcosa che non serve al Paese, che diffonderà disorientamento, che avrà un connotato totalmente devastante per il nostro sistema giudiziario, perché saranno processabili gli immigrati clandestini e gli italiani che sono i loro datori di lavoro.

Se non si fanno gli accordi internazionali, non si potranno rispedire a casa queste persone. Così si risolve il problema, non con le chiacchiere! In questo modo voi state facendo un danno al Paese, che ci costerà centinaia di milioni di euro e creerà

- la massa di soggiornanti irregolari, celebrando i processi con i costi che vi ho elencato, senza ottenere alcun effetto. Ci pentiremo, il Senato si pentirà di ciò che sta votando questa sera!

Questo per una questione squisitamente formale, in quanto la differenza di voti era ininfluente, ma per una questione di principio e di rispetto della regolarità del voto, questa Presidenza dispone che si torni a votare l'emendamento 19.108 a scrutinio segreto.

dell'avvocatura, considerato che si stabilisce che l'unica misura applicabile nei confronti degli accusati di determinati reati è quella della custodia cautelare in carcere. Il nostro sistema processuale processuale è impostato nel senso di ritenere la misura cautelare in carcere una misura residuale rispetto alle altre. Con la modifica che si propone, invece, si capovolge questo principio: la misura cautelare diventa la misura principale e le altre misure diventano misure residuali. Attualmente questo era possibile esclusivamente per i reati di mafia, mentre oggi si estende a una gran quantità di reati. Indubbiamente è una scelta difficile quella che ci apprestiamo a fare, me ne rendo conto, perché è un problema dibattuto da tantissimi anni. Però, penso che la situazione del nostro Paese, senza che questa voglia apparire una norma eccezionale, vada nella direzione

quella custodiale in carcere, certo nella speranza che le misure vengano adottate sulla base di elementi ponderati, valutati, verificati. La sfida di questa norma che si vuole introdurre, di questo capovolgimento del sistema sta proprio in questo.

a quei criteri che il giudice deve adottare nell'applicare la misura. Noi riteniamo che, tra gli elementi da valutarsi nell'applicare la misura, debba essere presa in considerazione la banca dati prevista dall'articolo 97 delle norme di attuazione, ossia la banca dati delle misure cautelari eseguite, ossia già pendenti ed eseguite nei confronti di un soggetto nuovo destinatario della misura.

estende questa innovazione, che privilegia la misura cautelare in carcere come misura prioritaria, a determinati reati per noi ugualmente gravi e non presi in considerazione. Si tratta di estendere questa misura al furto in abitazione

nel nostro Paese alcuni anni fa e che peraltro continua a verificarsi? Tre anni fa si parlò in modo particolare del fenomeno degli incendi dolosi che provocarono anche vittime. Non è pensabile che per un tipo di reato di questa gravità non possa essere prevista la misura cautelare in carcere. Per queste ragioni noi crediamo in questa norma che ci è stata proposta e vogliamo anzi rafforzarla attraverso i nostri emendamenti. Non illustro l'emendamento 23.0.100 perché è un emendamento particolarmente tecnico. In ogni modo,

nel senso che, qualora l'appello venga accolto, la misura cautelare deve essere eseguita.

Signor Presidente, faccio riferimento all'emendamento 23.103 perché forse, nella stesura del testo, il redattore del disegno di legge è incorso in un *lapsus calami* o in una svista nel coordinamento delle norme. Ricordo che qui si tratta sostanzialmente dell'articolo 275 del codice di procedura penale, che fa riferimento alla custodia cautelare in carcere obbligatoria, quindi nella sostanza a quella che una volta si chiamava il mandato di cattura obbligatorio. Questa situazione era ed è soprattutto prevista con le norme vigenti per i delitti distrettuali, realmente espressivi di una pericolosità sociale. In particolare quelli di terrorismo, sequestro di persona, traffico di stupefacenti, sfruttamento sessuale del minore ed altri ancora. Vengono esclusi con la normativa vigente quei reati che sono di minore rilevanza e gravità sociale, quali ad esempio quelli di natura informatica. Con la norma che si intende e che si vorrebbe introdurre e approvare in questo momento diventerebbe obbligatoria la custodia cautelare in carcere anche per quei reati

Va rilevato che per questi reati, che non sono espressivi di una particolare pericolosità sociale, si ritiene irragionevole estendere l'istituto dell'obbligatorietà della custodia cautelare. Ricordo come siano intervenute in materia sia la Corte costituzionale che la Corte europea dei diritti dell'uomo per sostenere che l'obbligatorietà della misura cautelare va limitata soltanto ai delitti che destano un grave allarme sociale e, in particolare, vengono citati i delitti di mafia. È evidente che estendere la custodia cautelare obbligatoria anche a reati quali quelli informatici, attribuiti alle procure distrettuali, non certo per la gravità ma per mere esigenze di coordinamento delle indagini, contrasta con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nonché con l'articolo 6 della Corte europea dei diritti dell'uomo sul giusto e corretto processo. Sarebbe pertanto censurata una tale norma certamente sia dalla Corte costituzionale italiana che dalla Corte di Strasburgo.